Onorevoli colleghi, il 21 ottobre scorso si è spento, all'età di 94 anni, Giuliano Vassalli. La sua esperienza di giurista, che si fonde pienamente con la sua vita politica e con l'attività sociale e istituzionale, comincia negli intensi anni di lotta nella Resistenza, per poi raggiungere il suo punto più alto nella nomina a giudice costituzionale e nella presidenza della Consulta. Giuliano Vassalli, uomo di diritto e professore, si è sempre distinto per l'ispirazione scientifica e per la sua fertile azione come uomo delle istituzioni, capacità preziose che emergono dalla sua costanza nel tradurre in azione politica, in atto legislativo, in decisione giurisprudenziale un'immensa e composita cultura che spaziava dalla criminologia al diritto processuale, dal diritto internazionale a quello comparato. Oltre alla coraggiosa militanza antifascista e all'attività parlamentare, l'eredità del professor Vassalli consiste proprio nella sua esperienza di giurista umanista, al servizio sia dei progetti di riforma della legge penale, sia di quei casi delicati che si presentavano frequenti nella realtà sociale italiana. Entrambi questi aspetti lo videro protagonista di un fondamentale rapporto fra scienza giuridica e società civile. Senatore della Repubblica nella IX legislatura, dopo l'elezione a Presidente della Commissione giustizia, diventa Capogruppo del PSI. In seguito, viene nominato Ministro della giustizia nel Governo Goria del 1987, nel Governo De Mita del 1988 e, ancora, nel VI Governo Andreotti del 1989. Quale Ministro di grazia e giustizia porta a compimento decisive riforme legislative, tra cui non si può non ricordare la stesura del codice di procedura penale e dei relativi correttivi, la disciplina del patrocinio gratuito per i non abbienti, la riforma della legislazione antimafia. In seguito, nominato giudice costituzionale, diviene Presidente della Corte nel 1999. Illuminante, sul metodo d'indagine giuridica da lui seguito e proposto, è la sua celebre frase: «Il diritto penale sostanziale, a onta della tensione umana che in ogni tempo lo percorre, è da millenni più o meno lo stesso. Per lo meno, nonostante i rivolgimenti storici, sono quasi sempre gli stessi - e limitati - i suoi problemi specifici: l'illecito, la colpa, la sanzione, la pericolosità dell'agente». Questa frase non inganni, tuttavia, perché la figura del professor Vassalli ha saputo dare voce forte, autorevole e convincente al miglior riformismo giuridico di questo Paese. Pochi uomini hanno avuto la stessa capacità di incidere sul tessuto normativo fondamentale: l'impianto accusatorio del nuovo codice di procedura penale, le necessarie correzioni alle asperità e alle contraddizioni del codice Rocco, il temperamento del sistema delle misure di sicurezza, fondato sulla pericolosità sociale, l'interpretazione insieme garantista e rigorosa delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario e delle misure di prevenzione. Questa è 1'immensa e ricca eredità che ci lascia il militante politico, 1'avvocato, il parlamentare, il ministro, il giudice, il presidente della Corte costituzionale Credo che per ricordarne il ruolo valgano le parole che egli stesso usò per descrivere la figura di Aldo Moro, suo amico e collega, meno di due anni fa, in occasione di un convegno commemorativo: «In lui era, sin dall'inizio, una duplice personalità di grande politico e di studioso di straordinario rilievo scientifico; insieme convivevano l'intensa attività politica e l'insegnamento universitario». Parole che accomunano, nel rimpianto e nel ricordo, due indimenticabili figure della nostra storia repubblicana.

va interpretato e va collocato nella storia del nostro Paese attraverso la sua intensa biografia. Penso che sia l'italiano illustre che più ha inciso attraverso diversi momenti del suo impegno. È stato politico e legislatore: politico attivo nella Resistenza (organizzò la liberazione di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat); politico quando venne arrestato e detenuto a via Tasso e torturato; politico quando fu consigliere comunale per il Partito socialista a Roma; politico quando fu deputato; politico quando fu senatore. Fu giurista e accademico, avvocato insigne e grande professore universitario. Componente di tutte le commissioni ministeriali per la riforma del codice penale e del codice di procedura penale sin dal 1946. Fu un insigne esponente dell'Esecutivo: Ministro della giustizia, ininterrottamente, sia pure in tre diversi Governi, dal 28 luglio

giudice costituzionale e Presidente della Corte. Ricordiamo che nella sua attività da Ministro, nel 1987, presentò il disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale, che vide poi la luce nel 1988 e, sempre nel 1987, fu suo il disegno di legge per la modifica del codice di procedura civile approvato nel 1990. Sempre nel 1990 insediò la commissione Pagliaro per la riforma del codice penale e per la produzione di un disegno di legge delega per la riforma del diritto sostanziale. Questi quattro momenti Giuliano Vassalli politico, Giuliano Vassalli uomo di governo, Giuliano Vassalli componente e presidente dell'organo di garanzia costituzionale, Giuliano Vassalli espressione dell'Esecutivo sono tutte tappe uniche di una coerenza scientifica e politica invidiabile. Noi lo ricordiamo, ma per farlo dovutamente è nostro dovere anche attualizzare il suo ricordo. Egli, come ci rammenta Mauro Ferri, fu inflessibile difensore dell'obbligatorietà dell'azione penale, cui collegava l'autonomia

come Mauro Ferri ha ricordato nella sua ultima visita fattagli il 12 ottobre, ossia nove giorni prima della sua morte: egli era amareggiato perché vedeva l'Italia in decadenza e regredita. Noi faremmo il nostro dovere di legislatori se ricordassimo questi Padri della Patria, il loro pensiero, la loro testimonianza, il loro impegno, la loro lungimirante visione delle cose. Facciamone tesoro: è l'unico modo per onorare i grandi italiani.

al cordoglio espresso in quest'Aula per la scomparsa del professor Giuliano Vassalli, un padre nobile di questa Repubblica e un insigne maestro. Giuliano Vassalli nacque il 25 aprile 1915, ed in questa data di nascita era già scritto parte del suo destino: diventò uno dei capi più autorevoli della Resistenza, di quella Resistenza fatta di lotta per la liberazione, ma soprattutto di rischi per la propria vita. Giuliano Vassalli ha ricoperto nella sua lunga carriera i più alti incarichi in ambito accademico e culturale, nonché in ambito politico e istituzionale. Non è mia intenzione ripercorrere, neppure per sommi capi, l'evoluzione della sua carriera accademica, culminata nell'attribuzione del ruolo di professore emerito di diritto penale presso l'università di Roma "La Sapienza". Mi basti dire che Giuliano Vassalli può a buon diritto essere collocato accanto ai grandi maestri del diritto, accanto a Carnelutti, Antolisei, Nuvolone, Leone e Pisapia, ovvero ai grandi maestri della scienza del diritto processuale penale. Si dice che la forza di una scienza è tanto più grande quanto più essa viene insegnata dai maestri e propagata a generazioni di allievi: Giuliano Vassalli nel suo insegnamento diede forza e vigore alla scienza del diritto processuale penale. La sua carriera in ambito politico e istituzionale fu altrettanto intensa: deputato, senatore, Presidente della Commissione giustizia del Senato, Ministro di grazia e giustizia, due volte candidato alla Presidenza della Repubblica, giudice della Corte costituzionale e suo Presidente. Fu Ministro dal luglio 1987 al gennaio 1991, in una stagione di incertezze e di ansie irrisolte; in quel ruolo fu il padre del nuovo codice di procedura penale, non a caso definito unanimemente codice Vassalli (il primo codice della Repubblica). La sua fermezza come Guardasigilli, che negando ogni proroga indusse il Parlamento e la commissione ministeriale al rispetto dei tempi tecnici che a molti erano parsi troppo brevi, portò un contributo determinante alla nascita del nuovo codice che sostituì, con una rivoluzione copernicana, il codice Rocco del 1930. da Guardasigilli affrontò il terreno incerto delle riforme, traducendo in norme i valori contenuti nei principi della nostra Costituzione, nelle sentenze della Corte e nelle Carte dei diritti dell'uomo. Inoltre, dimostrò che il processo penale è il prodotto di una determinata cultura, di un qualcosa che sta al di fuori e al di là del diritto. La procedura penale dà a quei valori extragiuridici concretezza operativa e potenza pratica e, senza quei valori di fondo, la procedura degenera in formalismo, viene neutralizzata e distorta a fini di parte. Vogliamo ricordarlo non solo per il rigore intellettuale e morale che lo caratterizzava, ma anche per l'impegno e la passione politica dimostrata all'interno delle istituzioni. Ebbi modo di leggere i suoi saggi, ma soprattutto ciò che mi colpì maggiormente furono le sue interviste riportate sui giornali. Un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera» nel 2003 rimase una pietra miliare per farmi comprendere esattamente ciò che poi è accaduto in questi ultimi anni. Sullo scontro con i magistrati Giuliano Vassalli disse: «È uno scontro epocale e istituzionale che si ripete. Epocale perché la Costituzione scritta dopo il fascismo volle rendere assolutamente debole il Presidente del Consiglio e forte e indipendente la magistratura. Istituzionale perché con la nascita del CSM nel 1958 si è creato un corpo separato con protezione costituzionale. Il Ministro» - concludeva Vassalli con un tono amaro in quella intervista - «viene considerato dai magistrati come un servo o un antagonista». Viviamo tempi difficili e convulsi che per ciò stesso dimostrano una scarsa vocazione per nuovi codici, vale a dire per rinnovamenti condotti secondo criteri sistematici. Ma l'opera di Giuliano Vassalli ci sprona nel cammino delle riforme affinché nel quadrante del processo penale le lancette riprendano a muoversi in senso orario, verso un sistema di tipo accusatorio nel quale sia escluso che l'imputato

che nel 2000 il professor Giuliano Vassalli donò alla nostra biblioteca la straordinaria collezione di opere di diritto comune e canonico edite nei secoli dal XVI al XIX appartenute al padre, Filippo Vassalli, anch'egli insigne e insuperabile maestro del diritto, in Opere che oggi sono esposte nella Sala Vassalli, al secondo piano del Palazzo della Minerva. Una munifica donazione fatta da Giuliano Vassalli con la stessa discrezione che lo ha caratterizzato sempre e segno di una grande affezione per lo straordinario patrimonio librario posseduto dalla nostra biblioteca.

Signor Presidente, con la scomparsa di Giuliano Vassalli l'Italia ha perso uno degli ultimi grandi campioni di quella straordinaria borghesia illuminata che ha dato tanto lustro alla storia politica e alla democrazia della nostra Repubblica. In anni lontani ho avuto il privilegio e l'onore di incontrare ripetutamente Giuliano Vassalli, di stringergli la mano, di ascoltarlo ed anche di conversare con lui su questioni serie. Ho un ricordo nitido di quegli incontri, come sempre succede quando avviciniamo personalità di straordinario spessore intellettuale. Di Giuliano Vassalli ho viva la memoria degli occhi vivacissimi, ironici e curiosi, della figura elegante, della precisione del linguaggio, dell'acutezza del ragionamento e della profondità delle intuizioni.

quest'Aula ha potuto meditare sullo straordinario coraggio, sino alla prova della tortura, con cui ha combattuto la guerra di liberazione nazionale, sul suo contributo al governo del Paese, all'azione del suo partito politico, al lavoro accademico e alla professione forense. Vassalli ha avuto come punto di riferimento costante in tutta la sua vita pubblica e istituzionale la Costituzione repubblicana. Ed è partendo dalla Costituzione che io leggo la sua lunga battaglia per l'introduzione del "giusto processo" nelle aule dei nostri tribunali, per garantire la parità tra accusa e difesa di fronte a un giudice terzo e imparziale. Sarà un Parlamento a maggioranza di centrosinistra - negli anni di un Governo di centrosinistra - a modificare l'articolo 111 della Costituzione, così introducendo il giusto processo nel nostro ordinamento. Colpisce, presidente Schifani, ricordare il bel garantismo di Vassalli oggi in quest'Aula, poco prima che un suo successore a via Arenula sia chiamato ad informare il Senato della Repubblica sulla morte orrenda di un giovane, Stefano Cucchi, entrato vivo, con le sue gambe, in un carcere italiano e, nel breve volgere di una manciata di giorni, uscito morto in circostanze misteriose ed equivoche. Oggi, qui in Senato, in un'Aula dove tante volte Giuliano Vassalli ha preso la parola, di lui si ricorda soprattutto la grande figura pubblica. La coerenza delle posizioni politiche, la fede socialista, l'amicizia con uomini del livello di Nenni e Saragat, la sapienza di uomo di diritto, la preziosa opera alla Corte costituzionale. Ma è alla personalità e allo stile intellettuale e morale di Giuliano Vassalli che dobbiamo anche guardare se vogliamo rendergli un onore pieno e completo. L'Italia d'oggi avrebbe grande bisogno di esempi di vita come Giuliano Vassalli. Era un uomo riservato ed integro, di forte impegno civile e di assoluta moralità. Equilibrato, scrupoloso, spirito autonomo e schivo, ha vissuto agli antipodi del carrierismo e del rampantismo che pure erano già tanto di moda anche nei tempi del suo impegno pubblico. Uomo politico e dirigente coerente del Partito socialista italiano, non conosceva cosa fosse il settarismo e coltivava una saggezza laica, sempre rispettosa dei valori di chi la pensava diversamente da lui. A noi che sediamo in Parlamento può essere di insegnamento ricordare come Giuliano Vassalli amasse le battaglie delle idee e detestasse la lotta tra le persone, come sapesse proteggere la sua vita personale con grande riserbo e riservatezza, come fosse nemico della personalizzazione in politica, come sapesse rivestire cariche pubbliche di grande rilevanza sempre con la modestia e il decoro che sono propri delle grandi personalità. La scomparsa di Giuliano Vassalli, signor Presidente, dovrebbe farci riflettere a fondo sulla condizione attuale del nostro Paese e su quanto sia cambiata, certo non in meglio, l'Italia d'oggi, dove emergono e prevalgono personalità tanto diverse da lui e e di tanto minore nobiltà civile. Avremmo molto bisogno nella nostra vita pubblica del buon esempio di esistenze specchiate come quella di Giuliano Vassalli, ma abbiamo quotidianamente davanti soprattutto cattivi modelli che arrivano a fare del decoro e della compostezza dei disvalori. Credo che in questa in questa pesante mutazione negativa della società politica italiana, che ci priva di punti di riferimento ideali e morali, stia tanta parte della crisi che l'Italia sta attraversando e tanta parte delle difficoltà di fondo che ancora ci impediscono di uscirne fuori. Le doti umane di Giuliano Vassalli, la sua profonda cultura e l'assoluta correttezza intellettuale di tutta la sua vita non sono valori prepolitici, né elementi secondari della sua personalità. Anzi, sostanziano un modo e uno stile di fare politica che oggi sono minoritari nel nostro Paese, ma che sono stati il dato distintivo di quegli uomini che, come Giuliano Vassalli, hanno fatto l'Italia democratica.

ricordare Giuliano Vassalli significa rendere omaggio a una inestinguibile fonte di autentica passione per la giustizia, che neppure la morte potrà essiccare. Scorrendo le oltre 4.000 pagine della raccolta dei suoi scritti, si percepisce la dimensione dell'opera, che spazia, come lei ha evidenziato, signor Presidente, dal diritto penale sostanziale alla procedura penale, dalla politica criminale alla criminologia. A Vassalli, inoltre, si deve il più significativo sforzo di riforma del sistema penale del dopoguerra: il Codice di procedura penale e il progetto di legge delega per un nuovo Codice penale

Se si vuole rintracciare un filo rosso di questa immane produzione, è al rapporto tra diritto e giustizia che ci si dovrà rivolgere. Laddove i due concetti paiono esprimere a volte valori confliggenti, allorquando situazioni storico-politiche li pongono in antitesi, ma anche quando, più prosaicamente, esigenze di certezza e ragioni di giustizia tendono a creare tra loro un contrasto. Si tratta insomma del tema del «diritto ingiusto», che apre nella coscienza del giurista una crisi che egli non può e non deve sfuggire. Ed è qui che l'insegnamento di Giuliano Vassalli si fa ininterrotta lezione etica. In questo solco possono essere collocati alcuni veri e propri classici del diritto che a lui si devono. Tra questi, «Limiti del divieto di analogia in materia penale», nel quale si indagano le barriere di garanzia poste a presidio della libertà del cittadino rispetto alle norme incriminatrici; «La potestà punitiva», forse la sua opera più importante, in cui ci si cala nel cuore del diritto penale per scoprire l'essenza del rapporto Stato-cittadino che esso suppone e definisce al tempo stesso. Da questi studi più lontani nel tempo, seguendo quel filo rosso, si risale fino alla recente opera dedicata alla punizione dei delitti di Stato nella Germania post-nazista e nella Germania postcomunista. Qui si ripercorre criticamente il travaglio della dottrina e della giurisprudenza tedesche - dopo il crollo del nazismo e poi del regime comunista della Germania Est di fronte al dilemma del valore da attribuire al diritto (anche penale) dei vecchi regimi, tanto più rispetto a comportamenti "criminali" che, perpetrati nella sua vigenza, da esso erano legittimati. All'esito dell'indagine Vassalli ci offre, oltre l'analisi storica, una ricostruzione generale che mira ad anteporre la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo quei princìpi previi che rimandano all'esistenza di un diritto naturale valido in ogni contesto e a dispetto di ogni regime - alla mera attuazione in chiave positivista delle normative del tempo. Giuliano Vassalli fu anche un politico. Approcciò la politica senza rinunciare al distacco dello studioso. Ma non fu mai un tecnico. Ebbe generosità e cuore per farsi uomo di parte e seppe non rinnegare la sua parte. lo fece quando da giovane antifascista fu incarcerato, torturato dalle SS e salvato *in extremis* dalla morte per intercessione di Pio XII. Non lo fece da senatore socialista, quando la bufera giudiziaria pretese di spazzare via quella esperienza politica. Fino in fondo è stato fedele alla sue passioni e alla sua storia, senza però restarne mai soggiogato. Seppe, semmai, dall'alto della sua saggezza, ricondurle nell'alveo della vicenda interrotta di una Nazione in cammino, in grado di superare i tanti drammi che ne hanno segnato la pur giovane esistenza. In tal senso mi piace ricordare l'onore che Vassalli volle fare al Senato accettando di introdurre il volume dei discorsi parlamentari di Alfredo Rocco, del quale era stato studente e allievo. Non era compito facile per chi aveva provato sulla propria pelle la durezza del regime di cui il maestro era stato esponente di primo piano. Ma Vassalli, nel cimentarsi nell'impresa, seppe tener conto di ciò che vi era di contingente nell'opera di Rocco e di ciò che invece ha acquisito valore nella durata. Ha criticato le norme condizionate dall'ideologia dello Stato autoritario sopravvissute alle riforme successive al 1944 e alla nuova Costituzione, ma con grande onestà intellettuale ha salvato quelle norme che si riconducevano al garantismo di tradizione liberale: stretta legalità delle norme incriminatrici e irretroattività delle stesse. Anche in questo caso restò fedele alla sua storia ma seppe pure indagare oltre, per scoprire qualcosa di ciò che ha unificato la Nazione e lo Stato oltre le stagioni, oltre i regimi, oltre le ideologie. Seppe discernere ciò che resta da ciò che è destinato a scorrere, come solo i grandi saggi sanno fare. Un esempio per tutti alla vigilia del centocinquantesimo anniversario della nostra Patria. Un invito a non omettere per timore di essere sconvenienti o politicamente scorretti.

(ha voluto esequie con pochi amici), ma la sua impronta, l'impronta che ha lasciato nella storia del nostro Paese, è invero, come tutti hanno ricordato, profonda ed ampia. Sono Sono condivisibili soprattutto quelle considerazioni che ci conducono - penso legittimamente - a ritenere Giuliano Vassalli uno dei Padri della Patria,

del quale ha condiviso fino all'estinzione, fino in fondo, le scelte. figura viene unanimemente riconosciuta e rispettata anche perché - come ha detto il senatore Zanda - era certamente un nemico della personalizzazione politica

di principi che potranno aiutare l'ulteriore attività di riforma di questo Parlamento con riferimento all'obiettivo di un processo effettivamente giusto. I suoi principi di riferimento consideravano soprattutto i diritti della difesa e le garanzie del cittadino. Penso che quelle sue intuizioni possano essere oggi ulteriormente riprese e considerate per un'attività di riforma che, ovviamente, non possiamo che auspicare quanto più condivisa. Nei prossimi giorni avremo modo di ricordarlo ulteriormente in un'aula messa a disposizione dal Presidente del Senato nel contesto del palazzo

poco fa, e che danno luogo ad un segmento importante della biblioteca del Senato. Lo ricorderemo Lo ricorderemo soprattutto con riferimento alla sua militanza nel Partito socialista italiano, al quale mi onoro di essere anch'io appartenuto e, grazie a quella comune militanza, porto in queste considerazioni un'emozione legata ai tanti momenti che abbiamo condiviso insieme nel partito e nelle attività parlamentari.

Si tratta di situazioni nelle quali un'inerzia nella nostra legislazione comporterebbe delle sanzioni a livello delle Comunità europee e della Corte di giustizia.

La principale di queste misure non è un adempimento ad una norma specifica europea, ma un adeguamento importante in un settore molto delicato che riguarda i servizi pubblici locali. A questo è dedicato l'articolo 15. Si tratta di una riforma che è stata tentata più volte nel passato e che con questo provvedimento giunge a realizzazione, rendendo maggiormente competitivo tale settore, con benefici per i cittadini, nonché per le municipalità e gli altri enti territoriali, cui potranno giungere risorse dalla cessione - in parte o per intero - delle quote di queste società.

misure per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche, finalizzate specificamente alla protezione dell'ambiente e segnatamente alla riduzione delle emissioni. L'articolo 5 si riferisce poi

dichiarazioni vanno però comunque acquisite e in questo articolo si individua il modo per poterlo fare sin dall'anno corrente. ad eliminare possibili incertezze interpretative che l'attuale formulazione della normativa circa l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari può ingenerare. contiene norme per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi.

altre norme in materia di controlli sulla sicurezza alimentare. Gli articoli 10, 11 e 12 disposizioni volte ad equiparare a tutti gli effetti le aziende che hanno sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea con quelle con sede invece nella Repubblica italiana. L'articolo 13 reca modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati, al fine di risolvere una procedura d'infrazione in

Dell'articolo 15 ho riferito in precedenza. All'articolo 16 ci sono norme particolarmente importanti a difesa del marchio "*made in Italy"* e dei prodotti interamente italiani per garantire che la qualità, la buona fama dei nostri prodotti non sia usurpata da un uso troppo facile di denominazioni, che possono indurre a credere che questi prodotti siano davvero espressione davvero espressione dell'apparato produttivo del nostro Paese. All'articolo 17 sono contenute norme sul sesto Censimento generale dell'agricoltura, indispensabile per poter, sulla base dello stesso, adempiere ad obblighi europei. All'articolo 18 vi sono disposizioni in materia di prelievo mensile. Infine, l'articolo 19 prevede norme riguardanti il recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, volte all'attuazione della decisione della Commissione europea sul

riguarda gli affidamenti della gestione di farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali.

nel corso dell'esame presso la 1a Commissione, un po' scherzosamente, nei dibattiti che si svolgono spesso in maniera informale, quello in oggetto è stato variamente ribattezzato come decreto «mille pseudo-infrazioni»

anche se va dato merito - parzialmente almeno - al presidente Vizzini ed al relatore Malan del fatto che, senza lo scrutinio, in alcuni casi rigoroso, da loro esercitato nei confronti di pressioni della maggioranza,

da un decreto in esame al Senato un emendamento non gradito al Quirinale, che avrebbe reso il Cavaliere meno esposto agli umori della magistratura, affermandosi anche che ciò avrebbe leso la sovranità del Parlamento.

la questione delle norme eterogenee, nonché prive dei requisiti di necessità ed urgenza. Faccio un solo esempio, che poi solleva anche problemi politici che esamineremo in sede di merito:

in sede referente alla Commissione politiche dell'Unione europea perché c'era una norma chiave sui servizi pubblici locali di cui non si poteva espropriare la 1a Commissione. 1a Commissione. Il problema è che quella norma non ci doveva proprio stare in questo decreto, perché non è attinente ad una infrazione. Avendo inserito una norma eterogenea abbiamo anche svuotato la Commissione competente del suo ruolo. Inviterei tutti i colleghi a leggersi anzitutto la presentazione che il Governo medesimo fa dell'articolo 15, dove si ammette che le sanzioni non ci sono. Si dice infatti che l'articolo 15 sta in questo provvedimento al fine prioritario di adeguamento all'ordinamento comunitario, non di introdurre Con questo argomento - «adeguamento dell'ordinamento comunitario» - si può inserire qualsiasi norma dentro un decreto del genere, svuotando, a parte gli strumenti ordinari, soprattutto la legge comunitaria, che avrebbe questo precipuo ruolo.

dalla collega Contini, approvato dalla maggioranza con l'astensione dell'opposizione, afferma chiaramente, nella parte motivazionale, che il provvedimento reca misure che non rispondono direttamente al criterio dell'urgenza proprio dello strumento del decreto-legge; inoltre, sul punto specifico dell'articolo 15, ricorda che c'è una delega aperta con la legge comunitaria 2008, e che ben si sarebbe fatto a procedere nel senso dell'attuazione di quella delega, e invitando a valutare l'opportunità di stralciare dal

consente infatti di adottare provvedimenti anche urgenti, ma nei confronti di obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso. È stato fatto un uso da cavallo di Troia di questo articolo della legge Buttiglione per motivi che non sono utilizzabili strettamente secondo la logica di quella legge che ha un valore ordinamentale. La pregiudiziale ricorda poi puntualmente gli emendamenti che non c'entrano con specifiche procedure di infrazione: si va dalla Guardia costiera alle concessioni autostradali, elettrodomestici e motori elettrici agli impianti portuali per i rifiuti, materie legate agli obblighi comunitari, ma non a scadenze obbligatorie immediate. Per di più, quand'anche ci trovassimo di fronte a scadenze cui far fronte immediatamente che richiedessero una soluzione univoca, per così dire in rime obbligate, ci sarebbe, nel nostro ordinamento, la possibilità di ricorrere alle Commissioni in sede deliberante, anziché necessariamente a decreti,

il primo è quello relativo alla eterogeneità del contenuto ed il secondo è quello della mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza che devono assistere la decretazione. Non possiamo omettere di ricordare che la legge n. 400 del 1988 all'articolo 15 stabilisce che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, così come non possiamo omettere di ricordare che con la sentenza n. 171 del 2007 la Corte costituzionale è intervenuta in materia di decretazione di urgenza riaffermando la necessità di una verifica puntuale e rigorosa dei presupposti di cui all'articolo 77, ossia i casi straordinari di necessità ed urgenza. L'articolazione della nostra questione pregiudiziale è ovviamente tecnica.

che contraddistinguono questa legislatura. È evidente una sorta di insofferenza da parte del Governo per il Parlamento, per il lavoro parlamentare, per cui il ricorso alla forma della decretazione non ossequiosa delle caratteristiche proprie dell'omogeneità, dell'urgenza e della necessità diviene il modo per bypassare il lavoro parlamentare. In una logica che ritiene appesantimento democratico la nostra funzione, peraltro duplicata attraverso le critiche ormai diffuse al bicameralismo perfetto, non solo

Riteniamo che la filosofia di fondo che accompagna la produzione legislativa del Governo nasconda nasconda una visione autoritaria dell'Esecutivo, una non fiducia nella centralità dell'istituto Parlamento, per cui dobbiamo provvedere ad esaminare i provvedimenti che il Governo licenzia, rinunziando alla nostra attività di iniziativa privandoci del nostro ruolo. È una realtà che i disegni di legge di iniziativa parlamentare vivacchiano o dormono nelle Commissioni, mentre le corsie preferenziali facilitano gli atti d'iniziativa governativa. Ancor più vengono agevolati gli atti di iniziativa governativa come quello come quello stiamo esaminando, ossia la decretazione d'urgenza, quando di urgente non vi è nulla e nulla è di straordinaria necessità. Dobbiamo riappropriarci del principio sacro della centralità del Parlamento. Non dobbiamo consentire che questo andazzo diventi norma vivente, perché attraverso la norma vivente dell'esproprio del Parlamento si determina la morte della democrazia parlamentare: esattamente il contrario del diritto vivente. Per questo motivo e per le ragioni tecnicamente esposte nella questione pregiudiziale QP2, essenzialmente riferentesi ai difetti dei presupposti di omogeneità,

Innanzitutto, per quanto riguarda la critica generale del collega Li Gotti circa la cosiddetta espropriazione del Parlamento, posso convenire che vi siano tanti, troppi provvedimenti governativi, ma devo anche dire che il Parlamento non è mai stato privato

La logica di questo provvedimento è di intervenire con urgenza su alcuni settori che lo richiedono in materia comunitaria: infatti, si parla di adempimento di obblighi comunitari nel senso ampio del termine e di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia, con ciò richiamando due ampi concetti riguardanti il diritto costituzionale europeo, secondo il quale, da una parte, vi sono procedure di preinfrazione e poi di infrazione, a norma dell'articolo 226, poi vi sono eventualmente procedure sempre di predeterminazione della pena ed eventualmente, tramite l'intervento della Corte, lo lo stabilimento e l'indicazione di queste sanzioni e pene. Tutto quello che riguarda il procedimento,

preinfrazione, certamente quando addirittura vi sia stata una sentenza della Corte di giustizia. Dico cose note a tutti, ma che è bene ricordare: allora, pur a fronte di una legge comunitaria approvata alla Camera, che dovrà essere discussa al Senato, gli articoli di questo provvedimento anticipano soluzioni per le ragioni di necessità e urgenza delle quali sto parlando.

o meglio lo fa, ma implicitamente - delle ragioni di particolare urgenza che coinvolgono alcuni di questi articoli, anche se si tratta

Si dice anche che mancano alcune logiche giuridiche

Tuttavia, non è stato ricordato che una successiva e fondamentale sentenza della Corte costituzionale in qualche modo torna indietro rispetto a quella del 2007, lasciando più spazio al legislatore e non andando a interferire se non nel senso di un'ampia coerenza del provvedimento. Credo che, ricordando il titolo del provvedimento - «Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee»

necessità, l'urgenza, la coerenza di materia e ciò che in qualche modo è sempre stato evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nella questione

delle Regioni con riguardo a determinati dati economici. Credo invece che, essendo la materia di competenza esclusiva dello Stato, Stato, qualche accenno a competenze diverse non comporti l'intervento *ex lege* delle Regioni, perché questi aspetti sono del tutto marginali la legge italiana si conforma agli obblighi comunitari mettendo in essere un sistema congruo e perfetto.

se vogliamo simpatica, ma assolutamente non aderente alla realtà del provvedimento stesso. Non entro poi nelle citazioni del quotidiano «il Giornale»,

Chiedo pertanto ai colleghi, ma mi permetto di chiederlo anche alle opposizioni, *re melius perpensa*, di rigettare le questioni pregiudiziali

dissentendo dalle considerazioni appena svolte dal collega (anche di Commissione) Boscetto,

ai rapporti Governo-Parlamento e tra maggioranza e opposizione, che vedono emergere posizioni anche molto diverse all'interno della stessa maggioranza relativamente

questo avrebbe un senso Chi non è interessato alla discussione è pregato quindi di lasciare l'Aula. ADAMO norme non pertinenti con il contesto, a cui sono state aggiunte, sia nella fase di esame in Commissione che con gli ultimi emendamenti presentati in Aula dal Governo e dal relatore,

porta avanti la privatizzazione dell'acqua in Italia senza regole particolari, come se si trattasse di un servizio qualsiasi e non di un bene essenziale e pubblico per definizione. Non

per non citare il famoso detto che a pensar male si fa peccato, ma si indovina - sembra proprio che questo ritardo sia voluto per permettere all'Aula, tramite un decreto-legge che ufficialmente dovrebbe occuparsi di procedure di infrazione che prevedono

che risulta davvero retorico, propagandistico e stucchevolmente falso il continuo richiamo alla presunta indisponibilità dell'opposizione al dialogo e alla collaborazione istituzionale.

la 1a Commissione aveva già iniziato a istruire i testi di legge depositati in materia e nominato i relatori, di maggioranza e di minoranza.

che le procedure d'esame di un testo di legge sono completamente diverse da quelle di un decreto, ed è per questo che siamo di fronte ad un esproprio, non perché non se ne possa

la tutela della vita privata. Nell'unico caso, Ministro, in cui l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea avrebbe dovuto essere assolutamente stringente e rigoroso, la proposta di emendamento tende invece ad una proroga, per cui gli utenti italiani, se passerà questo emendamento, saranno ancora disturbati in casa loro, al telefono

ai Comuni e che si sono tradotti in servizi, strade e quant'altro, dunque non in capitali all'estero da far rientrare con lo scudo fiscale, ma in servizi ai cittadini. Il Governo non ha combattuto abbastanza davanti all'Unione europea

della ricchezza patrimoniale di questi Comuni. Rischiamo non di vendere le quote azionarie delle società, ma di svenderle. E a vantaggio di chi, è ovvio; a svantaggio di chi, è chiarissimo: dei Comuni e dei cittadini che in quegli stessi Comuni abitano e hanno diritto ai servizi. Se questo è il federalismo fiscale che hanno in mente gli amici delle Lega e quelli della maggioranza, ritengo sia un fatto da spiegare molto bene a tutti gli elettori del Nord. *(IdV)*. Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, il decreto-legge n. 135 del 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, contiene norme eterogenee ed articoli in evidente contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, anche in merito alla decretazione d'urgenza. Mentre dovrebbe entrare in vigore l'agognato federalismo fiscale - agognato almeno per la Lega - alcuni provvedimenti della maggioranza e del Governo marciano contro il decentramento delle funzioni economiche ed amministrative e contro la stessa interpretazione della Corte costituzionale, che definisce la tutela della concorrenza non solo in senso statico, ma anche in quella accezione dinamica ben nota al diritto comunitario. È proprio la mancanza di concorrenza e la tutela che questo Governo e questa maggioranza offrono ed assicurano a monopolisti, oligopolisti e cartelli vari, con i quali vanno a braccetto e dai quali prendono ordini, come è dimostrato con lo svuotamento ed il rinvio della *class action* (sostituta dalla «*farce action»*, ossia una vera farsa, quella presa in giro degli utenti e dei consumatori ideata dal ministro Brunetta nei confronti della pubblica amministrazione, che non prevede alcuna sanzione ed alcun risarcimento dei danni che la burocrazia spesso infligge ai cittadini e alle famiglie) da determinare prezzi e tariffe molto più elevate della media europea e comunque di quei Paesi che applicano le corrette regole della concorrenza e del mercato nei diversi settori, dal gas all'energia, dai servizi bancari a quelli assicurativi.

che dovrebbe calmierare l'esosità delle banche ed offrire ai consumatori costi più contenuti e certezza nei tempi di accredito delle somme trasferite, oppure nel settore dei carburanti. In quest'ultimo una recente indagine di Federconsumatori e Adusbef, che ha messo a confronto i prezzi del gasolio del riscaldamento nei primi giorni di ottobre, ha confermato per l'Italia il triste primato del costo più alto al netto delle tasse locali, attestandosi al 9 per cento in più rispetto alla media europea e ben al 13 per cento in più rispetto alla Spagna. Tale differenza è ancora più marcata ed è pari al 41 per cento per chi consuma in media 1.000 litri di gasolio. Invece di incidere sulle cause che determinano stangate quotidiane sui consumatori e sulle famiglie liberalizzando quei settori, come il mercato del gas quasi insensibile alle regole della concorrenza - mi auguro che il monopolista ENI, mediante la sua controllata SNAM Rete Gas, non rafforzi la sua posizione dominante sul mercato acquistando E.On., in vendita in queste ore, ma lasci spazio ai competitori minori Governo e maggioranza vanno a liberalizzare con questa legge due settori: l'acqua, che è un bene comune per l'umanità, e le molestie telefoniche. Voi liberalizzate le molestie telefoniche! Non basta che alcune multinazionali del nostro continente siano detentrici di buona parte dell'acqua commercializzata nel mondo e che tante fasce di popolazioni tra le più povere nel mondo debbano sottostare al ricatto economico per non morire di sete. Questo decreto, se convertito in legge, sottrarrà ai cittadini e alla sovranità delle Regioni e dei Comuni - cari amici della Lega, cari senatori della Lega l'acqua potabile del rubinetto, il bene più prezioso, per consegnarlo a partire dal 2011 agli interessi delle grandi multinazionali e farne un nuovo *business* per i privati. Noi dell'Italia dei Valori pensiamo che sia un epilogo da scongiurare, sia per un concetto inviolabile che annovera l'acqua come diritto universale e non come merce da immettere nel mercato, ma anche per le ripercussioni disastrose che una privatizzazione potrebbe generare sui cittadini in funzione

che nella giornata di martedì 20 ottobre, con una delibera di Giunta regionale, ha sancito l'avvio della ripubblicizzazione dell'Acquedotto Pugliese,

Le molestie telefoniche sono previste e regolate dall'ordinamento in quanto costituiscono il reato di cui all'articolo 660 del codice penale, se fatte per petulanza o altro biasimevole motivo con l'effetto di arrecare al destinatario disturbo. Con l'approvazione dell'emendamento Malan - voglio ricordare che c'è stata già una proroga di un anno con il famigerato emendamento Fleres - si offre alle aziende la possibilità di usare, per la propria attività promozionale, le banche dati tratte dai vecchi elenchi telefonici (precedenti (precedenti all'agosto del 2005). Paradossalmente, in questo modo, anche coloro che esasperati dalle assillanti e moleste campagne telefoniche avevano chiesto la cancellazione dagli elenchi pubblici, saranno di nuovo bersaglio del *marketing* telefonico. Questo Governo ci tiene tanto alle famiglie che non le vuole lasciare tranquille neanche all'ora di pranzo o di cena, perché con l'approvazione di questo articolo, in deroga alla legge sulla *privacy*, ogni cittadino può essere molestato con offerte di servizi tra i più vari. Questo è un Governo che l'unica cosa che sa liberalizzare sono le molestie! Mentre su altri settori le liberalizzazioni marciano con forte ritardo. Questo emendamento va contro gli interessi e i diritti fondamentali dei cittadini e, cosa estremamente grave, si scontra con i provvedimenti già presi a tale proposito dal Garante per la protezione dei dati personali, secondo il quale le operazioni di «*teleselling*» potevano avvenire solo sulla base di banche dati regolarizzate, in cui tutti gli utenti interessati avevano espressamente fornito il consenso al trattamento dei propri dati per scopi pubblicitari (con la possibilità, tra l'altro, di revocare tale volontà in qualsiasi momento). Qualsiasi civiltà giuridica - non sono un giurista, ma lo dico ai Presidenti di Commissione e ai tanti giuristi

lo debba richiedere espressamente; non che alcuni servizi molesti vengano appioppati alla generalità delle famiglie e che occorra disdettarli se indesiderati. Signor Presidente, concludo perché so che fra qualche minuto il Ministro riferirà su un altro fatto di gravissima rilevanza, dicendo che questo emendamento è una mostruosità giuridica da parte di una maggioranza molesta, che liberalizza le molestie telefoniche riducendo le famiglie a merce di scambio con i desiderata delle aziende. Per questo, noi dell'Italia dei Valori, faremo tutto il possibile per evitare l'approvazione della liberalizzazione del bene comune acqua e delle molestie telefoniche.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la seguente informativa muove da una premessa:

Ecco perché il Governo è in prima linea nell'accertamento della verità. Ecco perché sentiamo per intero il dovere di impegnare tutte le nostre energie per accertare chi, con qualsiasi comportamento commissivo ovvero omissivo, ha determinato questo tragico quanto inaccettabile evento. Per fare ciò il Governo si è immediatamente attivato acquisendo le informazioni che erano prontamente disponibili; nei diversi ambiti istituzionali sono stata già avviati i necessari controlli e ci si è impegnati per acquisire al più presto tutti i risultati. dunque, venendo nello specifico al tema dell'informativa, segnalo che, alle ore 23,30 circa del giorno 15 ottobre 2009, Stefano Cucchi è stato tratto in arresto da alcuni militari della stazione dei carabinieri Roma-Appia per rispondere del reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riferito dal Ministero delle difesa, la fase dell'arresto e quella della successiva perquisizione si sono svolte senza concitazione e senza particolari contatti fisici, dal momento che il fermato si trovava in condizioni fisiche particolarmente debilitate e si era dimostrato intenzionato a giustificare la propria posizione giudiziaria piuttosto che a contestarla. Peraltro, Stefano Cucchi, anche durante la perquisizione domiciliare avvenuta in presenza della sua mamma, era apparso preoccupato dalle reazioni della famiglia, oltre che dalle eventuali conseguenze penali che sarebbero seguite al suo arresto per droga. Quindi, aveva mostrato immediatamente un atteggiamento collaborante. Durante la permanenza presso i locali della stazione carabinieri Appia, e più precisamente dalle ore 23,40 del 15 ottobre alle ore 3,30 circa del 16 ottobre, risulta che il Cucchi è stato custodito e guardato a vista dagli operanti e successivamente accompagnato presso le camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Tor Sapienza, ove è stato preso in carico alle ore 3,55. Qui Stefano Cucchi è stato trovato lucido, cosciente ed in condizioni di salute compatibili con lo stato di detenzione, senza ferite o ecchimosi diverse da quelle tipiche della tossicodipendenza in fase avanzata. Intorno alle ore 5, Stefano Cucchi ha contattato con il campanello il piantone della camera di sicurezza, dichiarando di soffrire di epilessia e manifestando un generale stato di malessere. Dalla documentazione acquisita dal competente Ministero della difesa risulta che, pur contro la volontà dell'arrestato, è stato richiesto l'intervento di personale del «118» e che all'arrivo dei sanitari Cucchi ha rifiutato sia di sottoporsi a visita, sia di essere accompagnato presso una struttura ospedaliera. Ciò nonostante, è stato disposto l'accesso del sanitario nella camera di sicurezza per consentire il controllo visivo dell'arrestato e per procedere alla redazione delle previste certificazioni sanitarie, nelle quali si è dato atto della volontà di Stefano Cucchi di non ricorrere ad un ricovero ospedaliero. Alle ore 9,20 circa del 16 ottobre, Stefano Cucchi è stato condotto presso il tribunale di Roma per la convalida dell'arresto. In attesa della celebrazione del giudizio con il rito direttissimo è stato poi affidato al personale della polizia penitenziaria per la detenzione nelle camere di sicurezza del Palazzo di giustizia. Alle ore 12,30 circa, Stefano Cucchi è stato accompagnato dai carabinieri presso le aule dibattimentali. Prima dell'inizio del giudizio Stefano Cucchi ha potuto incontrare il padre, con il quale si è intrattenuto a parlare in totale autonomia ma vigilato a distanza. Durante l'intera udienza, durata circa mezz'ora, non è stata riferita né rilevata nessuna anomalia, tant'è che l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto ed ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendola dunque compatibile con lo stato di salute dell'imputato. Immediatamente dopo, alle ore 13,30 circa, Stefano Cucchi è stato nuovamente preso in consegna dal personale della polizia penitenziaria, dopo le usuali operazioni di passaggio di responsabilità certificate da documentazione in cui, sul piano delle condizioni fisiche, nulla viene rilevato di anormale o incompatibile con la detenzione. ore 14,05, Stefano Cucchi è stato refertato dal medico dell'ambulatorio della città giudiziaria, il quale ha riscontrato «lesioni ecchimotiche in regione palpebrale inferiore bilateralmente» ed ha avuto riferite da Stefano Cucchi medesimo lesioni alla regione sacrale ed agli arti inferiori, queste ultime non verificate dal sanitario a causa del rifiuto di ispezione espresso dal detenuto. Condotto al carcere di Regina Coeli, Stefano Cucchi è stato regolarmente sottoposto a visita medico di primo ingresso. Il referto clinico redatto dal medico di guardia dell'ambulatorio dell'istituto ha evidenziato la presenza di «ecchimosi sacrale coccigea; tumefazione del volto bilaterale orbitaria; algìa della deambulazione degli arti inferiori». Il medico, inoltre, ha dato atto di quanto riferito da Stefano Cucchi medesimo, e cioè di un senso di nausea e di astenia e di una caduta accidentale dalle scale necessitante, a parere dello stesso sanitario, di esami RX cranio e *videat* neurologico regione sacrale e di visita ambulatoriale urgente presso ospedale esterno. Alle ore 19,50 dello stesso giorno, Cucchi è stato accompagnato con autoambulanza all'ospedale Fatebenefratelli, dove è giunto alle ore 20,01. Visitato presso la predetta struttura ospedaliera, a Stefano Cucchi sono state riscontrate la frattura corpo vertebrale L3 sull'emisoma sinistro e la frattura della vertebra coccigea. Sebbene invitato al ricovero, Stefano Cucchi ha rifiutato l'ospedalizzazione ed alle ore 22,31 è stato quindi dimesso con 25 giorni di prognosi e contro il parere dei sanitari. Tradotto nuovamente a Regina Coeli, Stefano Cucchi è stato ricoverato per osservazione presso il locale centro clinico diagnostico-terapeutico e collocato in stanza detentiva con altri tre detenuti. Il giorno 17 ottobre, Stefano Cucchi, che lamentava nausea e dolenzie diffuse, è stato nuovamente visitato dal medico dell'istituto penitenziario, il quale, riscontrati quelli che il detenuto riferiva essere i postumi di una caduta accidentale, ha evidenziato una lieve dolorabilità alla palpazione profonda dell'addome e dolenzia speciale in regione sacro-iliaca ed ha disposto ulteriori accertamenti da effettuarsi presso il Fatebenefratelli. Trasferito nella struttura ospedaliera, dove giunge alle ore 13,25 del 17 ottobre, Stefano Cucchi ha richiesto il ricovero in ospedale a causa del persistente dolore della zona traumatizzata e per riferita anuria. La diagnosi fatta dai medici dell'ospedale è stata la medesima del giorno precedente. Alle ore 19,45, sempre del 17 ottobre, il Cucchi è stato ricoverato presso il reparto di medicina protetta dell'ospedale Sandro Pertini, dove è deceduto tra le ore 6,15 e le ore 6,45 del 22 ottobre, del 22 ottobre, da certificazione medica risultante dal certificato rilasciato dal sanitario ospedaliero, per presunta morte naturale. Secondo quanto riferito dal Ministero della salute e delle politiche sociali, il paziente Stefano Cucchi è giunto in reparto in barella e con l'indicazione dello specialista ortopedico a non assumere posizione eretta. Il paziente era portatore inoltre di catetere vescicale posizionato dai medici dell'ospedale Fatebenefratelli per il controllo della diuresi. All'esame obiettivo il medico della struttura di medicina penitenziaria ha riscontrato ecchimosi in sede palpebrale superiore ed inferiore bilaterale. Tali lesioni, come spiegato dallo stesso Cucchi, sarebbero state riportate in conseguenza ad una sua caduta avvenuta accidentalmente il giorno prima del suo compleanno. Gli esami radiografici effettuati hanno confermato la presenza delle fratture già diagnosticate dai sanitari dell'ospedale Fatebenefratelli a carico della colonna vertebrale. Giova evidenziare che proprio nel corso della visita medica il Cucchi ha ribadito verbalmente quanto già sottoscritto all'atto dell'ingresso in reparto, e cioè il non consenso alla diffusione di notizie sanitarie a chiunque, inclusi i suoi familiari. Tale posizione di chiusura nei confronti dell'esterno è stata peraltro confermata all'infermiera del reparto dallo stesso paziente la domenica pomeriggio. Il Cucchi, sempre secondo quanto comunicato dal Ministero della salute, è stato sottoposto quotidianamente a visita medica internistica e all'effettuazione di esami di laboratorio. Inoltre, è stato visitato per due volte dal consulente ortopedico. Durante il ricovero il paziente ha mantenuto un atteggiamento scarsamente collaborativo, rifiutando - secondo quanto riferito dai sanitari - la visita oculistica ed alcuni accertamenti radiografici ulteriori. Relativamente alle condizioni generali, il Ministero della salute ha riferito che il Cucchi era in condizioni di magrezza estrema. Lo stesso ha mantenuto durante il ricovero una alimentazione spontanea ed ha continuato a bere, anche se in quantità ridotte; ha rifiutato la somministrazione per via endovenosa di liquidi e sostanze nutrienti; inoltre, l'apporto idrico e calorico è stato potenziato - così risulta nel diario infermieristico - attraverso l'assunzione per bocca di succhi di frutta. «La morte purtroppo» - recita il virgolettato dei sanitari - «è sopraggiunta in maniera improvvisa ed inaspettata». Il paziente, secondo quanto dichiarato dai sanitari, «si è mantenuto sempre lucido ed è stato in grado di decidere, manifestando ora il consenso, ora il diniego alle cure ed agli accertamenti diagnostici e specialistici». «I medici» - riferisce sempre il Ministero della salute - «hanno deontologicamente rispettato la volontà del paziente». Passando ad un piano più squisitamente amministrativo, rappresento che sin dal 23 ottobre 2009, e cioè sin dal giorno dopo la morte di Stefano Cucchi, con provvedimento della competente Direzione generale dell'Amministrazione penitenziaria è stata affidata al provveditore regionale del Lazio una indagine immediatamente avviata e volta ad appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto. Tempestiva altrettanto è stata l'indagine penale avviata dal procuratore di Roma, con la quale indagine il giorno dell'avvenuto decesso ha provveduto ad iscrivere il relativo fascicolo al n. 8047/09 ed ha incaricato il consulente tecnico di turno di effettuare un esame autoptico della salma del Cucchi, assicurandosi che i prossimi congiunti del defunto avessero ricevuto avviso dei propri diritti e facoltà. L'incarico peritale è stato espletato in data 23 ottobre del 2009 alla presenza del consulente tecnico di parte nominato nel frattempo dai familiari della persona deceduta, assieme ad un altro consulente. Al riguardo, comunico che proprio ieri l'ufficio di procura ha esteso l'incarico peritale ad un collegio di consulenti d'ufficio incaricandoli, in accordo con i consulenti di parte, di effettuare ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla salma del detenuto e sulla documentazione medica acquisita. In attesa degli esiti della consulenza peritale, la procura ha comunque avviato ogni attività di indagine utile alla completa ricostruzione dei fatti e all'accertamento delle cause della morte. pur non essendo io a conoscenza di questioni inerenti il segreto istruttorio, posso comunicare all'Assemblea, in base a quel principio di leale collaborazione che lega il Ministro agli uffici giudiziari, che due sono i grandi filoni dell'indagine che sta conoscendo

Inoltre, necessita un chiarimento riguardo ai mancati colloqui tra Stefano Cucchi e i suoi familiari. Le notizie che mi sono state comunicate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e che sono state acquisite dalla stessa direzione della casa circondariale di Rebibbia riferiscono che i familiari di Stefano Cucchi si sono presentati alle ore 22,30 di sabato 17 ottobre e alle ore 12,30 di lunedì 19 ottobre presso il reparto di medicina protetta dell'ospedale Sandro Pertini per avere un colloquio con il proprio congiunto. In entrambe le occasioni ai familiari di Stefano Cucchi è stata rappresentata la necessità di fornirsi preventivamente, come la legge prevede, di un permesso di colloquio per essere legittimati all'incontro. Quanto alla richiesta dei genitori di Stefano Cucchi di parlare con i medici della struttura ed al diniego loro opposto di incontrare i sanitari, rappresento - così come l'Amministrazione penitenziaria riferisce - che nel caso specifico si è data applicazione all'accordo esistente con la ASL di Roma, che prevede che nessuna informazione, a nessun a nessun titolo, venga data ai parenti e/o aventi diritto senza esplicita e formale autorizzazione da parte della magistratura competente. Questo divieto può essere superato in presenza di un'autorizzazione del detenuto a rilasciare notizie mediche ai familiari. Tuttavia, come si evince dalla documentazione, Stefano Cucchi non ha rilasciato alcuna autorizzazione in tal senso, manifestando per iscritto la propria volontà di non autorizzare i sanitari al rilascio di notizie mediche ai propri familiari. Questa la cronologia dei fatti sinora accertati. Rimaniamo tutti in attesa dell'esito, che vogliamo sia chiarificatore, degli ulteriori e complessi accertamenti medico‑legali e investigativi ancora in corso. Ma sia chiaro sin da ora che ai cittadini tutti e alla famiglia Cucchi in modo speciale dovrà essere al più presto fornito ogni dettaglio di verità, con la garanzia che gli eventuali responsabili dell'evento saranno chiamati ad assumersi le proprie responsabilità senza sconto alcuno.

i nostri sentimenti di condoglianze che non sono certamente rituali, ma sono rivolti con grande affetto perché è certamente incolmabile la perdita di un giovane di soli 31 anni, per il solo fatto che la morte di un giovane è già di per sé una grande ingiustizia. Vogliamo - come lei diceva Ministro, ma credo che lo vogliano tutti - chiarezza e verità. Il fatto è così grave da sembrare quasi estraneo a quello che è lo stato di diritto nel quale ci piacerebbe continuare a pensare che viviamo.

è bene aspettare l'esito delle stesse con grande fiducia, ma è bene anche continuare ad insistere sull'accertamento della verità, per un dovere primario che abbiamo nei riguardi della famiglia, ma anche nei riguardi delle istituzioni e di tutti noi che abbiamo il dovere di sapere e conoscere la verità fino

sulle immagini dei tanti soggetti che, a vario titolo, si trovano coinvolti in questa sconcertante vicenda: penso alle forze dell'ordine, alla polizia penitenziaria, ai medici e ai magistrati che non hanno concesso i domiciliari. Penso al fatto che sia stato negato ai familiari il permesso di parlare con i medici che curavano Stefano.

e anche a quelli che sono, più in generale, tutti i problemi che anche un caso come questo pone di fronte alle tematiche più grandi e ampie delle giustizia,

a vario titolo, abbia la tentazione di insabbiare nulla, ma che ciascuno voglia, con la delicatezza del caso, arrivare alla verità

in quest'Aula, non avrebbe mai dovuto aver luogo. Se però questa tragedia si è consumata ed è arrivata fin qui, mi conforta pensare che tutto questo possa avere un senso. Tutti noi, colleghi, colleghi, dobbiamo sentirci in dovere di chiedere che la verità sia certa e rapida e che la giustizia sia avvertita chiara, giusta e tangibile da parte delle vittime e del Paese:

al di là dell'umana compassione, constatare che in questo caso è lo Stato - e lo Stato di diritto - ad uscirne sconfitto: si è sconfitti quando viene tradito il dovere della sanità pubblica di curare e guarire; si è sconfitti quando viene infranto il dovere delle forze dell'ordine di proteggere e tutelare dalla violenza tutti, nessuno escluso; si è sconfitti quando viene ignorato il dovere del Governo di perseguire il bene pubblico di tutti i cittadini, che si realizza anche attraverso l'accertamento della verità; si è sconfitti quando lo stesso Governo, nella persona di un Ministro, assolve acriticamente alcuni membri di un'Arma senza che la giustizia abbia fatto il proprio doveroso corso. corso. Tutto ciò è stato commesso, signor Ministro, nei confronti di Stefano Cucchi: ecco perché sento il dovere di non porle tutte le domande che vorrei, che non vengono dalla lettura dei quotidiani, ma sono nate dalle mie personali visite in carcere e nelle caserme e dai quesiti che ho potuto rivolgere direttamente alle persone coinvolte in questi giorni. Ebbene, proprio perché ho toccato con mano e visto con i miei occhi la fine dello Stato di diritto, signor Ministro, io ed il mio partito sentiamo il dovere di leggerle non le nostre domande,

ai medici dell'ospedale dov'era ricoverato, che però si sono sottratti; alle guardie penitenziarie, ma le è stata chiusa la porta in faccia.

si dice: «Premesso che in un Paese civile e democratico come l'Italia non deve e non può succedere che un uomo venga consegnato sotto la tutela dello Stato in normali condizioni fisiche e psicologiche e dallo Stato venga poi restituito dopo soli sei giorni morto e in condizioni di un'atrocità disumana, in quali circostanze esatte mio fratello, Stefano Cucchi, si sarebbe procurato quelle molteplici lesioni? Perché la famiglia di Stefano ha saputo della sua morte solo ore dopo il suo decesso e soprattutto tramite il decreto del pubblico ministero di nomina del medico legale per l'autopsia? Perché viene dichiarato che Stefano era senza fissa dimora? Perché non è stato chiamato l'avvocato che Stefano aveva richiesto, assegnandogli invece l'avvocato d'ufficio? A Stefano, profondamente religioso, è stata data l'estrema unzione?». Queste domande non hanno avuto risposta per la famiglia. Ne seguono altre, di domande, che saranno oggetto di interrogazione parlamentare. Risponda lei, alla famiglia, a Ilaria che è qui presente, signor Ministro, e così facendo risponda a tutti i cittadini. Ci chiarisca una storia ancora oscura, e lo faccia non ripetendo la formula che ha usato il 27 ottobre - «una caduta accidentale» - perché non possiamo accettarla, signor Ministro; ma aiuti l'emergere della verità utilizzando ogni strumento a sua disposizione per il compiersi rapido di una giustizia che in Italia è stata veloce spesso solo per assolvere chi aveva potere e sempre lenta per condannare chi era protetto dal potere. La storia di Stefano è una storia fatta di orari che non tornano, come quello dell'arresto: è avvenuto alle ore 22, come si legge nel verbale di convalida dell'arresto inoltrato al tribunale, o alle ore 23,30 come sostengono i carabinieri? È una storia di lividi che appaiono sul viso, sul collo e dietro la nuca e che si vedono chiaramente nelle foto scattate all'arrivo di Stefano nel carcere di Regina Coeli, che io stesso ho visto con i miei occhi, ma che non c'erano quando lui è uscito di casa 18 ore prima. È una storia di malasanità, che assegna il codice verde, quello per le non urgenze, all'accettazione di Stefano in ospedale ed è poi costretta ad assegnare il "codice nero" all'uscita dall'ospedale cinque giorni dopo. Sono convinto che alla base di questo fallimento dello Stato ci sia la paura: la paura delle istituzioni nei confronti dei cittadini, tanto che vengono chiuse loro le porte, e la paura dei cittadini nei confronti delle istituzioni, che sempre più appaiono capaci di fare ciò che sono invece chiamate a contrastare. La paura, signor Ministro, nasce dall'ignoranza, e quindi solo con la verità la paura può essere dissipata. Ecco perché chiedo a lei, signor Ministro, di farsi carico che la verità giunga subito. Sono passati venti giorni. Ma la paura può essere fugata anche da leggi giuste: ecco perché chiedo a voi colleghi di impegnarvi per far sì che queste leggi giuste vengano introdotte nel nostro ordinamento. Penso alla legge che istituisce il reato di tortura e lo punisce severamente, non dovendo così obbligare la giustizia a procedere per omicidio preterintenzionale. anche ad una legge che permetta di superare le difficoltà burocratiche che si frappongono all'umano incontro tra famiglia e detenuto in condizioni critiche. Fino alle condanne definitive della magistratura non è in nostro potere né in nostro diritto esprimere dei giudizi su quanto compiuto da chi ne è responsabile. La giustizia deve fare il suo corso e per farlo velocemente non può venire delegittimata ogni giorno. La nostra condanna per ora si può limitare solo a quanto non è stato fatto, perché è chiaro che Stefano Cucchi è morto e ciò che doveva essere fatto dalle istituzioni che lo avevano in custodia ed in cura è stato disatteso. Ma si può morire così? In Italia si può morire di malattia, ma non si può morire di carcere o di malasanità! Ecco, allora, che mi chiedo e le chiedo: se scopo essenziale tra quelli dello Stato è assicurare l'incolumità ai cittadini, non certo agire per infrangere questo diritto, quello di Stefano Cucchi è ancora Stato, signor Ministro? La verità vera o la dite oggi o la cercheremo noi per Stefano e per tutti quelli che da oggi dubitano della verità non vera che sta uscendo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, abbiamo ascoltato con attenzione le sue parole, e ci tranquillizzano, perché abbiamo capito che c'è la determinazione e la volontà di approfondire questo increscioso episodio, sicuramente drammatico, che ci fa riflettere anche sul tema dell'afflittività della pena. Infatti, se non vogliamo essere ipocriti, sappiamo che il carcere ha una ineludibile funzione afflittiva: la pena è una pena e quindi porta anche ad una sofferenza psicologica. Su questo tema dobbiamo quindi riflettere, valutando attentamente se il regime carcerario odierno può essere corretto in alcuni aspetti, ma non facendo gli ipocriti e nascondendo che comunque l'istituzione carceraria ha un'ineludibile funzione afflittiva che rimarrà:

quindi dobbiamo trattare questa vicenda con attenzione, ma non dobbiamo dimenticare gli altri 147 casi che si sono verificati passando assolutamente sotto silenzio.

ci porta a ragionare sul fatto che la sofferenza psicologica e la rottura dell'equilibrio psicologico di una persona condotta in carcere possono portarla a compiere il gesto estremo:

La nostra è una situazione grave, ma non disperata, che va risolta all'interno dell'istituzione carceraria con interventi di controllo costante ed in questa direzione il Governo si è già mosso con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, vogliamo la verità

è dovuta a chi la chiede e - me lo lasci dire - anche all'Arma dei carabinieri, al Corpo della polizia penitenziaria e alla comunità dei medici italiani, che hanno il diritto di sapere chi di loro è stato infedele rispetto ai doveri che incombevano sul loro lavoro. Le chiedo di farsi garante, signor Ministro. Noi apprezziamo che lei sia qui sia qui e questo in qualche modo - mi lasci usare questa espressione - può essere considerato non solo un atto di rispetto

ho riflettuto non solo su come lo Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo di polizia penitenziaria, gli ospedali, i tribunali, i giudici, i medici sono intervenuti, ma su come alla cronistoria che lei ha fatto mancasse l'umano. Poc'anzi il collega Pedica ha detto che l'annuncio della morte di Stefano Cucchi è stato dato alla famiglia con la notifica del decreto con il quale venivano fissate la data e l'ora dell'autopsia. Ed io le chiedo, visto che lei è giurista e quindi conosce questa tensione inesausta che c'è sempre tra le regole di accertamento della verità, che sono stabilite dal codice e dalle garanzie, e la verità stessa, stavolta di farla, per se stesso e in nome nostro, tormentosa questa ricerca. Questa tensione deve essere un tormento. tormento. Dobbiamo sapere cosa è accaduto a Stefano Cucchi, e lo dobbiamo sapere per lui e per i tanti altri che cadono dalle scale e che, fortunatamente, non muoiono, di cui nessuna notizia e nessuna registrazione si hanno mai. A lei che è garantista, e lo è per formazione, per cultura politica e per proclamazione, le chiediamo di essere garantista fino in fondo e di cominciare ad essere garante degli ultimi. ultimi. Ciascuno di noi sa, infatti, come le vicende giudiziarie, le traduzioni, le detenzioni sono diverse se si è tra i primi o se si è tra gli ultimi, e sono gli ultimi che purtroppo affollano di più le nostre carceri. E magari ci spieghi com'è che Stefano Cucchi non aveva un avvocato di fiducia. E ci spieghi perché può capitare che il carcere sia per alcuni luogo di privilegio e per altri luogo di abbandono e di sopraffazione. E visto che lei è Ministro e aveva promesso un piano carceri che non abbiamo visto, la prego di farsi garante del fatto che bisogna andare in fondo alla faccenda e comprendere quanto sia un errore considerare la questione carceraria come un fatto di edilizia penitenziaria. È anche questo, perché la dignità è fatta anche di luoghi degni e magari, chissà, anche di circuiti alternativi per espiare le pene. Le chiedo di farsi carico, inoltre, dell'istituzione del Garante nazionale dei detenuti e le chiedo di capire se l'intercettazione casuale fatta a Teramo nasconda l'odioso, orrendo fatto isolato o se, in qualche modo, da questo si possa scendere a capire di più, a fare un affresco. Io non lo credo. non lo credo. Mi sono occupata di carceri per vent'anni nella mia vita e so come senza la polizia penitenziaria la riforma carceraria non avrebbe camminato. Però so anche che possono accadere cose orribili quando si è senza potere e si è ridotti nella privazione della libertà. Lei, che è Ministro della giustizia, si faccia garante di capire perché Diana Blefari può morire impiccata in carcere, perché i suicidi sono 17 volte di più in carcere di quanti siano fuori, perché c'è un sovraffollamento che non è figlio del caso e magari discende da certe scelte di politica criminale che introducono aggravanti o reati ideologici inefficaci sul fine della prevenzione e, magari, del controllo di un fenomeno come quello migratorio, ma che sono tanto simbolicamente efficaci. E dunque, che importa se le carceri arriveranno a 70.000 detenuti quando sì e no ne possono contenere dignitosamente 40.000? Insomma, signor Ministro, le chiediamo di farsi garante di tutto questo perché sta nella sua responsabilità e perché oggi lei è venuto a dirci che intende farlo.

GASPARRI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che la vicenda di Stefano Cucchi, che colpisce la sensibilità di tutti e ci sconvolge, non possa essere affrontata diversamente da come anche il ministro Alfano ha fatto poc'anzi in Aula, offrendo innanzitutto al Parlamento gli elementi puntuali che le varie amministrazioni - sanitaria, delle forze dell'ordine e della polizia penitenziaria - gli hanno fornito e concludendo in maniera chiara e facendosi già interprete nella sua premessa - che condividiamo che la verità va ricercata senza fare sconti a nessuno, in nessun ambito. Credo inoltre che l'immediatezza del suo intervento, la chiarezza delle sue parole e gli elementi che ci ha offerto siano quello che in questo momento il Senato

le autodifese gratuite che si sono sentite in questi giorni. La magistratura deve lavorare in modo sereno». Ecco, credo che questo atteggiamento dei familiari - la vicenda non è certo privata, è pubblica, tant'è che ne stiamo parlando in Parlamento, perché

determinazione nella ricerca della verità e di fiducia nella magistratura che, in ultima analisi, sarà quella che risponderà alle domande. Il Governo svolgerà le sue inchieste amministrative (le sta già facendo), il Parlamento discuterà, ma poi chi si pronuncerà, come è ovvio e come deve essere, sarà la magistratura.

sentito - cibo e acqua? E perché i medici non sono intervenuti? Possono intervenire? E si può forzosamente alimentare e idratare una persona? Sono tutte questioni sulle quali in altri contesti ci siamo interrogati e sulle quali tutti dovremmo riflettere, perché è strano

verità. Probabilmente non sarebbe morto, ma certamente la distruzione del fisico ha reso quel ragazzo ancora più debole ed esposto agli errori drammatici che

prioritaria. Siamo certi che il Governo, tutte le amministrazioni interessate - anche quelle sanitarie del Lazio - e la magistratura in ultima sede daranno le risposte alla domanda di verità che è di tutti noi in quest'Aula del Senato.

un ulteriore vuoto legislativo relativamente al decreto Amato del 2007, adottato all'indomani dell'omicidio Raciti in relazione all'accesso alle manifestazioni sportive. Il collega Benedetti Valentini ha presentato una proposta di legge in Commissione affari costituzionali che cerca in qualche modo di fare chiarezza in merito all'articolo 9 di quel decreto, facendo proprie e trasformandole in norma alcune delle interpretazioni date dall'Osservatorio

e pubblicata in data 29 luglio 2009, perché è assolutamente urgente conoscere le intenzioni del Governo circa il futuro dell'Antonio Merloni Spa e dell'economia del territorio della fascia appenninica, dove si trovano i relativi insediamenti. Ricordo che il 12 novembre scade il termine per i bandi di vendita dell'azienda commissariata e ancora non sembra vi siano manifestazioni di interesse in proposito. di ieri i lavoratori dell'azienda sono saliti sulla cima della torre di Nocera Umbra per manifestare preoccupazione circa il proprio futuro e per porre all'attenzione del Governo, delle istituzioni locali e nazionali il problema della loro azienda, chiedendo solleciti interventi in proposito. quindi, mettere in piedi entro breve un piano per una gestione condivisa della crisi aziendale tra le Regioni Umbria, Marche, Emilia Romagna e istituzioni statali attraverso l'attuazione della proposta di accordo di programma per sostenere l'occupazione e rilanciare la produttività dell'area. Al momento, le Regioni hanno dimostrato disponibilità in tal senso, sono pronte alla sottoscrizione, e nella mia interrogazione si chiedono le intenzioni del Governo circa volontà e tempi di sottoscrizione dell'accordo di programma quadro.